di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali,

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

nella seduta pomeridiana del giorno precedente è proseguito l'esame degli emendamenti e degli articoli fino all'articolo 24.

al comma 5, stabilisce che, nel giudizio sulla controversia promossa per ottenere la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in caso di pronuncia del giudice a favore del lavoratore, il datore di lavoro debba risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

come precisazioni. È in atto un'operazione di recupero di situazioni di contratto a termine irregolari, ma nei casi

volto a prevenire l'abuso della firma di dimissioni in bianco, ma quella legge è stata abrogata all'inizio di questa legislatura. L'emendamento 25.0.1 mira a risolvere lo stesso problema

ma consente a quest'ultimo di revocare l'eventuale atto falsificato dal datore di lavoro, senza bisogno di andare in giudizio e far valere - con le difficoltà che si possono immaginare - la falsificazione del documento.

di eliminare una piccola barbarie che sappiamo quanto sia diffusa tra le imprese meno scrupolose. Per questo motivo, chiediamo ai relatori, alla maggioranza e al Governo di valutare attentamente questo nostro emendamento.

delle indennità di disoccupazione legate all'effettiva ricerca di lavoro. Questo problema ormai si pone da molto tempo si propone di creare uno sportello unico per il lavoro. In tal modo, chi aiuta nella ricerca del lavoro e pretende che l'individuo si attivi è unito a chi paga le indennità;

i due enti, si può rendere più efficace il controllo sulla ricerca di lavoro e quindi rendere attivi e non assistenziali anche i sussidi.

che impone agli enti locali di progettare prioritariamente con gli uffici tecnici interni. Oggi, però, con la riduzione dell'incentivo dal 2 per cento, allo 0,5 per cento, ciò significa aver bloccato l'attività di progettazione interna degli enti locali. In un momento di grave difficoltà per il comparto delle autonomie locali, questa possibilità di progettare internamente rappresentava una valvola di sicurezza. Confidiamo, pertanto, nella ragionevolezza dell'Aula, dei relatori e del Governo sull'opportunità di reintrodurre questa percentuale. Essa arrivava fino al 2 per cento: non era necessario erogare il 2 per cento ma le amministrazioni potevano arrivare ad erogare fino al 2 per cento, con quella formulazione che prevedeva che il restante 1,5 per cento venisse versato su un apposito capitolo del bilancio dello Stato, è una formulazione a nostro avviso sbagliata, che sta creando grossi problemi e sta costringendo gli enti locali ad inventarsi delle forme di di accordi integrativi e di contrattazione decentrata per riuscire a rimpinguare questo 0,5 per cento, assolutamente troppo basso per consentire la progettazione interna degli enti locali. Davvero, quindi, noi confidiamo in una prova di ragionevolezza dell'intera Aula.

Presidente, questa è una norma di fondamentale importanza per riavviare una serie di attività, di lavori pubblici e di appalti, soprattutto negli enti pubblici. Condivido l'emendamento del senatore Mazzatorta, e ritengo che sia un incentivo alla realizzazione di progetti con i funzionari, con gli ingegneri e con i tecnici delle amministrazioni. Pur tuttavia, l'accoglimento di questo emendamento comporta un problema di copertura, perché il finanziamento è collegato a

tagliati nelle finanziarie e negli interventi anticrisi che si sono succeduti negli ultimi mesi e che sono davvero ridotti all'osso. Pertanto il nostro voto sarà di astensione.

Presidente, vorrei solo chiarire, per evitare che sorgano fraintendimenti su questo punto, che il fondo creato raccoglie l'1,5

i Comuni e le autonomie locali non versano questo 1,5 per cento nel bilancio dello Stato, altrimenti vi sarebbe una chiara lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Quindi, ad oggi, quel fondo non sta ricevendo nessun

Signor Presidente, vorrei dichiarare che mi asterrò dalla votazione su questo emendamento perché, se è vero che gli uffici tecnici delle amministrazioni locali hanno diritto al riconoscimento di un incentivo per la progettazione, è altresì vero che non può essere consentito a dismisura che ci sia un trattamento interno in netta contrapposizione con le libere professioni che limita in modo assoluto l'accesso al mercato. Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole a questo emendamento e vorrei far cadere un velo di ipocrisia che aleggia anche nelle dichiarazioni

atteso che gli enti locali non lo versano perché non hanno l'obbligo di farlo, con questo emendamento si ripristina una possibilità per gli enti locali di risparmiare sulla progettazione.

legge n. 443 del 1985 (legge quadro per l'artigianato), che è l'unica istituzione a cui si può fare riferimento per definire l'artigianalità e l'attività dell'impresa stessa.

quelle imprese che cessano l'attività o che comunque non risultano più in attività, si dice che sarà l'INPS, ente che da 20 anni è in contrasto con le commissioni provinciali per l'artigianato, proprio sul tema della decisione dell'artigianalità dell'impresa. Le commissioni provinciali infatti hanno titolarità nella decisione che l'INPS quasi sempre non riconosce;

infatti è anomala perché tale è la sua interposizione nel sistema dei rapporti giuridici tra l'albo delle imprese artigiane e l'INPS per quanto riguarda l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dei soggetti tenuti all'obbligo contributivo in materia previdenziale, con la conseguenza di dare nuovamente vita ad un conflitto di competenze ultraventennale in materia di potestà di iscrizione e cancellazione ai fini previdenziali delle imprese artigiane. La formulazione del testo legislativo risulta, come dicevo, ambigua a cominciare dalla finalità dichiarata, che sembra contrastare con quanto stabilisce il successivo testo del medesimo articolo, per continuare con la incomprensibile disposizione circa l'inopponibilità all'INPS delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto decorsi due anni dal verificarsi dei presupposti, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti iscritti alla gestione, soprattutto nelle fattispecie nelle quali non siano più ravvisabili i requisiti di qualifica artigiana in capo ad un soggetto e ad un'impresa ovvero nei casi in cui l'impresa stessa non sia più esistente. In tal modo, verrebbe violato il principio giuridico della corrispettività tra contributi e prestazioni, poiché, mentre da una parte vi sarebbe l'obbligo, legislativamente imposto dall'articolo in esame, di versare i contributi anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano più dovuti, dall'altra si verificherebbe l'effetto perverso di non poter erogare le correlative prestazioni previdenziali e pensionistiche, poiché mancherebbe il requisito della prestazione dell'attività lavorativa. Per questo chiediamo di sopprimere l'articolo. *relatore*. Signor Presidente, mi sembrano interessanti le osservazioni formulate

accettare una riformulazione nella quale sia prevista l'inopponibilità all'INPS decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, ma anche sentite

vorrei fare qualche riflessione su tale vicenda, anche perché è stata oggetto di grandi commenti da parte dei giornali, e poi suggerire una soluzione, sulla quale peraltro ho discusso a lungo anche con i colleghi.

Signor Presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta su questo emendamento perché una sovracopertura, ossia una copertura evidentemente eccedente. È del tutto chiaro che, essendoci una copertura eccedente, per quel che concerne il profilo di finanza pubblica il parere non può che essere di nulla osta. però, è stato sempre connesso, per prassi, ad una richiesta: ove l'emendamento con maxi copertura fosse stato approvato dalla Commissione,

Naturalmente alla Commissione bilancio ciò non è sufficiente, perché avremmo bisogno di un'asseverazione da parte del Tesoro. formulare un parere favorevole all'emendamento, quindi alla soppressione della copertura, in quanto una puntuale disamina del caso porta ad affermare che l'onere o è insussistente come sembra dalla relazione dell'INPS - o al massimo potrebbe essere trascurabile. Pertanto, signor Presidente, dopo aver discusso con i colleghi e data la particolarità del caso che è stato già dibattuto all'interno dell'Aula, ritengo di poter esprimere parere favorevole all'emendamento, ai sensi dell'articolo 100, e quindi di dare un nulla osta allo stesso,

questa asseverazione venga prodotta in termini corretti sulla scorta dell'INPS dal Tesoro, come nelle Commissioni bilancio. In conclusione, signor Presidente, ribadisco il parere di nulla osta

bilancio. L'eliminazione della copertura non determina problemi rispetto alla sostanza dell'emendamento, che peraltro è stato discusso con

determinando poi le condizioni di tranquillità formale che il Presidente della Commissione bilancio ha ritenuto opportunamente di sottolineare esprimendo anche una valutazione positiva anche da parte dei membri dell'opposizione della Commissione bilancio.

il quale vuole tornare a lavorare; invece, in base alla nostra legge - che stiamo modificando con questa piccola misura - sarebbe obbligato ad andare in invalidità.

ma anche alla loro superiore attenzione, avendo loro per prime segnalato ciò di cui il relatore di maggioranza non si era avveduto; riconosco quindi una loro superiore qualità professionale. infatti, di novellare la norma del 2007 che prevedeva la scadenza dell'esercizio del diritto di delega a due anni, se non aumentassimo di 12 mesi la durata della delega ci troveremmo nella bizzarra condizione di avere la legge approvata

Con l'articolo 28 conferiamo una delega al Governo per attuare una riforma radicale e complessiva in senso universalistico degli ammortizzatori sociali.

si diceva sino a poco tempo fa - i migliori nel mondo. Poiché la delega al Governo richiede un lasso di tempo che può anche essere procrastinato sino a 24 mesi, questo emendamento si pone l'obiettivo di dare una risposta alla diffusa platea di lavoratori e famiglie privi di qualsiasi protezione sociale. Ora non abbiamo necessità di parlare dei parametri economici di ripresa che possono essere già avvistati, però una cosa è certa: anche su questo punto, siamo tutti d'accordo sul fatto che anche quando la ripresa - quantunque lenta e debole - riattiverà la nostra economia,

gli apprendisti hanno una protezione sociale di tre mesi, se hanno avuto modo di lavorare per un periodo equivalente. Certamente si tratta di misure frammentate,

migliora la copertura delle risorse economiche messe a disposizione degli ammortizzatori sociali, offrendo la possibilità che una quota almeno del 25 per cento delle maggiori entrate derivanti

quindi si tratterebbe di una ripresa economica molto lieve. Ma soprattutto essa non interverrebbe positivamente sul gravissimo problema dell'occupazione, che - insisto - permane. Abbiamo avuto un aumento di disoccupati pari a circa 500.000 unità nell'ultimo anno, e si prevede un aumento di disoccupati di circa di circa 1 milione per il 2010, anno che tutti prevedono sarà estremamente negativo su questo versante. Di qui la nostra insistenza per la riforma degli ammortizzatori sociali. Altro che una delega a 36 mesi!

rapporti di lavoro subordinato. Le risorse ci sono. Ribadiamo anche oggi che il fondo dell'INPS negli ultimi cinque anni ha registrato un

Sono presenti in tribuna gli studenti del «Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode» di Roma. Rivolgiamo loro il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio.

*(PD)*. Signora Presidente, ci ostiniamo a proporre i nostri emendamenti sul lavoro femminile, sulla conciliazione e sulla condivisione, a costo di apparire noiosi e pedanti,

caso dell'Answers di Pistoia. Comprendiamo la sfiducia di tante giovani donne che hanno studiato con successo, ma che restano fuori dal mercato del lavoro. E ancora, comprendiamo la frustrazione

Grazie, signora Presidente. Dicevo che comprendiamo anche la frustrazione di quel 20 per cento di donne che sono costrette a lasciare il posto di lavoro quando nasce il primo figlio e che non riescono a rientrare sul mercato del lavoro quando lo vorrebbero. Vogliamo dire alle donne italiane che non è per un destino cinico e baro che tutto questo accade, che misure più adeguate si potrebbero prendere, ma che non lo si vuole fare. Le nostre proposte partono da una realtà già molto negativa, che in altre occasioni abbiamo illustrato e che non ripeto qui. La crisi sta semplicemente aggravando una situazione negativa: indossiamo la maglia nera in Europa, 11 punti sotto la media europea. Per venire alle proposte, molto rapidamente ne citerò soltanto alcune. Proponiamo detrazioni o assegni per le lavoratrici madri come riconoscimento del lavoro di cura; un credito di imposta per le aziende del Sud che assumano donne; un sostegno all'imprenditoria femminile.

per le lavoratrici madri, la possibilità del *part time* con un periodo di contributi figurativi a carico dello Stato, ed altre misure che non ho tempo qui di illustrare. Prevediamo ancora, anche in questi emendamenti, il congedo paterno obbligatorio e la modifica della legge sui congedi parentali per renderli più convenienti anche per i padri, e quindi per gli uomini. A noi questa sembra una conquista di civiltà, nel nome, davvero, della condivisione del lavoro di di cura e delle responsabilità familiari.

per il mercato del lavoro, e quindi le politiche attive del lavoro e le riforme necessarie al sostegno della partecipazione delle donne al lavoro - il Governo di fatto non si vuole occupare. Ha lasciato scadere la delega;

compresa l'ex Italimpianti. Su questo c'è stato un grande impegno ‑ e a Genova glielo riconoscono tutti: maggioranza, opposizione e sindacati ‑ da parte del sottosegretario Viespoli, ma la situazione sta diventando davvero preoccupante

per consentire ai lavoratori di non veder messa in discussione la propria pensione in un momento in cui i posti di lavoro non ci sono più.

di attenzionare ‑ e mi auguro che l'ordine giorno sia focalizzato su questo punto ‑ il disagio sociale che rischia di determinarsi se non si interviene su una questione che è giusto affidare al corso che sta avendo, sul terreno amministrativo e non solo.

le attività di intermediazione devono essere effettuate solo da agenzie qualificate e strutturate. Non ci può essere un'attività di intermediazione "fai da te", come in qualche modo si ricava dall'insieme dell'articolo.

il termine «intermediazione» è estremamente vago nel suo contenuto, mentre l'espressione «attività di diffusione e scambio di informazioni» è molto più precisa e pertinente. quanto riguarda l'emendamento 28-*ter*.205, vorrei ricordare che l'unica vera questione essenziale è che questa attività sia svolta a titolo gratuito nei confronti del lavoratore.

C'è una norma dell'Organizzazione internazionale del lavoro che vieta che i servizi di collocamento, di intermediazione o di informazione nel mercato del lavoro siano resi a titolo oneroso nei confronti dei lavoratori. Vogliamo forse dire che è inammissibile la convenzione dell'OIL?

*Il Senato approva

*relatore*. Il tema è delicato. A fronte della presentazione da parte del Governo di un emendamento soppressivo, mi permetto sommessamente di chiedere una votazione per parti separate.

da parte del datore di lavoro della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 296 del 2006 abbia avuto luogo entro il 30 settembre del 2008.

Il relatore non ha chiesto il ritiro dell'emendamento 28-*octies*.200, ma una votazione per parti separate rispetto alla soppressione.

il relatore e il Governo sono al corrente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 399 del 5 dicembre 2008, ha ha stabilito che è incostituzionale vietare la prosecuzione delle collaborazioni continuative stipulate precedentemente all'entrata in vigore del decreto‑legislativo n. 276 del 2003.

Chiedo qual è il senso della sua soppressione, poiché mi è totalmente incomprensibile. Ho il testo della sentenza, nel caso il Governo non ne disponesse.

del relatore che è composto di due parti. Questo emendamento sopprime il comma 1 e riformula il comma 2.

insisto per chiedere che il relatore ci spieghi il significato, rispetto alla sentenza della Corte costituzionale, della soppressione del primo comma. infatti, capire quale sia l'intendimento di questo emendamento soppressivo, rispetto ad una sentenza della Corte costituzionale che ci vincola a fare il contrario.

tant'è vero che nella motivazione della prima formulazione del suo emendamento il relatore aveva preso le mosse proprio da una riflessione sull'effetto, forse non del tutto coerente con le intenzioni

l'assunzione a tempo indeterminato loro proposta per effetto dell'accordo sindacale successivo, hanno dimostrato disinteresse rispetto alla qualificazione rafforzata della loro relazione professionale, propongo una riformulazione che corrisponde al precedente

con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.".».

che lei, sottosegretario Viespoli, così attento a questo problema, non abbia potuto cogliere in quest'articolo una diminuzione della tensione della lotta a questo fenomeno, che riguarda

all'evasione e al lavoro nero mi pare sia un errore grave: per questa ragione voteremo contro e ci aspettiamo che il Governo riveda queste norme, che non ci fanno onore rispetto ad una piaga del nostro Paese.

i risultati e i numeri. In questo caso, però, ci troviamo di fronte ad un problema relativo alla esternalizzazione di alcuni servizi che, nel momento in cui sono stati esternalizzati, hanno determinato una copertura finanziaria per cinque anni. Quella copertura finanziaria non si è riproposta;

L'applicazione di tale coefficiente dovrà essere integrata e modulata alla luce del posizionamento comparativo di ciascuna amministrazione in termini di efficienza organizzativa e di produttività netta del fattore lavoro.

Presidente, assistiamo, attraverso ordini del giorno e talvolta emendamenti (che magari sono stati anche schivati per quanto riguarda questo provvedimento, ma non del tutto lo sono state alcune espressioni degli ordini del giorno), al tentativo di reintrodurre il tema del territorio come discriminante rispetto ad alcuni diritti fondamentali. Questo vale in generale: questo è stato il tema dell'accesso ai concorsi, proposto con un emendamento in cui si richiedeva all'accesso la residenza (norma assolutamente incostituzionale perché lo si può chiedere per la permanenza, ma non per l'accesso). Ritorna il tema della territorializzazione per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, ritorna il tema del coefficiente territoriale per quanto riguarda la contrattazione. Non siamo assolutamente favorevoli a questa impostazione, non perché non crediamo nella flessibilità, nelle specificità, nella possibilità di articolare diversamente le forme di contrattazione: ma tutto ciò non passa per una divisione del territorio con queste forme e in questi modi. Pertanto, anche su questo ordine del giorno esprimeremo il nostro voto nettamente contrario.

favorevoli ad un adeguamento territoriale degli stipendi, che corrisponde ad un sistema di equità: chiaramente contrari al sistema di gabbia territoriale definita come contrattazione nazionale diversificata, ma favorevoli se legata al secondo livello di contrattazione, che è proprio quello territoriale o d'area. Queste sono le posizioni dei sindacati e questa è la posizione che manterrà la Lega; e speriamo che l'Assemblea segua questo indirizzo.

ci si interpreta (cioè qualcuno interpreta la posizione di qualcun altro), che abbiamo sempre ritenuto, come Partito Democratico, che sia a livello di contrattazione decentrata che si deve tener conto delle specificità di produttività

così come non andava bene la formulazione rigida dei 70 anni di età. In questo modo, viene fatto salvo il principio dei 65 anni per il pensionamento per i medici e viene sanata una disuguaglianza tra medici ospedalieri e medici universitari, permettendo al singolo

questo emendamento permette al sanitario la scelta sulla propria età pensionabile: se mantenerla a 65 anni o se sfruttare la possibilità di arrivare fino a 70

adeguare la condizione di tutti i medici al privilegio che è stato concesso solo ai primari, in rincorsa a un ulteriore storico privilegio, appannaggio solo ed esclusivamente degli universitari e dei magistrati. Durante l'approvazione del cosiddetto primo decreto Brunetta, avevamo tutti congiuntamente presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo a rivedere il trattamento pensionistico dei sanitari, uniformandolo a quello delle altre funzioni pubbliche. Io ritengo che questo sia il metodo giusto. Con l'approvazione di questo emendamento andiamo a sanare una piccola parte di questa stortura, dando la possibilità anche ai non primari e ai non universitari di adeguarsi agli altri. La via maestra, però, continua a rimanere quella di togliere il privilegio ad altri (mi riferisco, ovviamente, alle baronie universitarie e della magistratura, che continuano ad averlo) e non quella di continuare una rincorsa nel tentativo di adeguare altri a quel privilegio.

per affrontare una disuguaglianza da eliminare. Certo, hanno ragione i colleghi che sostengono che forse questo non è il percorso ottimale: dovevamo partire dall'alto, riequilibrare tutto, forse abbassando il limite e concedendo ai giovani di essere immessi su un canale di lavoro importante. Oggi, però, noi concediamo a quei giovani di non essere rottamati, e questo è già un fatto importante. Su questa posizione, ritengo che tutto il Gruppo del PdL, ma anche altri colleghi che hanno espresso

soltanto per rilevare un profilo che a me pare di particolare interesse in questa norma.

Signor Presidente, nell'esprimere soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo

l'adozione e l'affido in Italia sono una materia molto delicata e difficile. È particolarmente difficile che vengano adottati o affidati bambini con handicap gravissimo,

che tipologia di attività possono fare e che non possono assolutamente ricevere compenso dai lavoratori, norma prevista dagli accordi internazionali. Mi pare non sussistano dubbi.

Potremmo dire, vista la lunghezza dei tempi che ha caratterizzato il provvedimento, che almeno di questo possiamo essere contenti. Tuttavia questo rimane per noi l'unico motivo di soddisfazione. In questi tre giorni di dibattito in Assemblea abbiamo sostanzialmente visto ripetersi un copione cui avevamo già assistito in Commissione: viene presentato il testo; si presentano gli emendamenti (magari all'ultimo minuto); grande e partecipato dibattito; grandi apprezzamenti per le utili osservazioni portate da ciascuno; ma poi, la maggioranza tira dritta per la sua strada, boccia tutti (o quasi) gli emendamenti dell'opposizione e fa sostanzialmente tutto da sola. Atteggiamento legittimo, per carità! La maggioranza governa (sottolineo che governa, non comanda). tutto ciò sarebbe maggiormente apprezzabile se le norme che costituiscono il risultato finale di questo lungo procedimento fossero, non dico totalmente condivisibili, ma almeno nella maggior parte apprezzabili.

il testo che ci accingiamo a votare è sostanzialmente quello uscito dall'esame delle Commissioni riunite 1a e 11a; un testo, sottolineo, che sino alle ultime due sedute delle Commissioni contava una ventina di articoli e che poi, tra il 29 ottobre e il 18 novembre, ha subito un vero proprio assalto, che lo ha trasformato in un mostro di oltre 50 articoli, sugli argomenti più disparati, ben lontani dal suo oggetto. Ma cerchiamo di illustrare più dettagliatamente quali sono i punti più critici del provvedimento, quelli che sono alla base del voto contrario che tra poco il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà su questo testo. Anzitutto lo spirito di fondo del provvedimento, che è stato ben illustrato dal collega Pardi in discussione generale: nella logica di un incontro libero delle forze del lavoro nell'ambito del mercato, lo Stato fa un passo indietro. se questo rafforzamento e valorizzazione dell'autonomia delle parti non fa i conti con la diversità delle parti stesse, se ciò si verifica su un terreno dove la bilancia delle forze è totalmente sperequata a favore dell'azienda, non si afferma un principio progressivo, che garantisca cioè la parte più debole, ovvero il lavoro e colui che fornisce il lavoro; abbiamo, invece, una situazione in cui l'azienda viene favorita proprio perché ha di fronte degli interlocutori deboli. Tutto ciò si è sostanziato nell'accantonamento o l'abbandono totale, già iniziato con il decreto-legge n. 112 del 2008, di tutte le innovazioni positive e condivise che erano state faticosamente raggiunte dal Governo Prodi con una trattativa democratica, aperta e costruttiva con le parti sociali, che si erano sostanziate nel protocollo sul *welfare* e nella conseguente legge n. 247 del 2007.

che io mi rifiuto di chiamare legge Biagi perché la considero un'offesa alla memoria e al pensiero di un bravo economista del lavoro, che ha comportato la proliferazione del morbo del precariato nel nostro mondo del lavoro: il ritorno alla somministrazione di lavoro a tempo determinato; l'attenuazione delle sanzioni contro il lavoro sommerso; le modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro; la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale; la nuova normativa in materia di aspettativa dei dipendenti pubblici; la norma limitativa sul riscatto dei congedi di maternità o parentali; la modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap. E, ancora, l'uso strumentale, come ha spiegato egregiamente il collega Treu, delle norme sulla certificazione del contratto di lavoro; per non parlare poi dell'introduzione, totalmente insensata, per mezzo dell'articolo 24, della riforma degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. A proposito di questo, è stato detto dal relatore che si tratta di una stratificazione normativa virtuosa; si è detto di approvarlo, e che poi nella pratica si vedrà. Due argomentazioni che a mio avviso - credo che colleghi ben più competenti di me condivideranno - sono la negazione di quello che un buon legislatore dovrebbe fare in una materia così delicata. La stratificazione normativa, con l'introduzione in un testo organico di norme scollegate dalle restanti parti del medesimo testo nel quale vengono inserite - stiamo parlando del codice di procedura civile - è quanto di più negativo si possa immaginare. Quanto poi alla seconda argomentazione, essa è il classico modo con cui il legislatore non si assume la responsabilità di adottare una posizione netta su una materia delicata, scaricando sulle spalle dei soggetti che saranno chiamati ad applicare la normativa - in questo caso la magistratura del lavoro - l'onere di dare loro l'esecuzione più consona, naturalmente riservandosi la possibilità di addossare poi a quegli stessi soggetti le responsabilità per gli eventuali malfunzionamenti della normativa. Vi è poi il problema delle deleghe al Governo per quanto concerne la disciplina in tema di lavori usuranti, sulla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del *welfare* e, cosa ancor più pericolosa (non naturalmente dal punto di vista procedurale, ma in base alla considerazione dello spirito con la quale ci si accinge ad affrontare la materia, esplicitato purtroppo dalle dichiarazioni di vari membri del Governo), sul riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Siamo sostanzialmente in presenza di deleghe in bianco che, considerate unitamente a quanto previsto dall'articolo 28, che rinvia ulteriormente l'esecuzione di quanto stabilito dalla legge n. 247 del 2007, significano l'espropriazione al Parlamento della sua funzione legislativa su materie di importanza capitale nell'attuale momento di crisi economica e sociale. Tutto ciò è davvero in contrasto con quanto stabilito in materia di delega legislativa al Governo dall'articolo 76 della Costituzione. Come ha detto il collega Li Gotti illustrando la questione pregiudiziale presentata dal nostro Gruppo, il Parlamento deve fare le leggi e non ratificare ciò che impone il Governo, sovente anche con il voto di fiducia. di legge n. 1167 - a pensare che l'unica delega per la quale il testo in esame dettava una serie almeno decente di parametri a cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nell'emanazione dei decreti delegati fosse quella sul diritto allo studio universitario contenuta nell'articolo 6-*bis*, dichiarato - giustamente, diciamo noi - inammissibile.

È qui necessario ribadire quanto già segnalato con la questione pregiudiziale: i disegni di legge collegati dovrebbero contenere interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria, in quanto funzionali alla realizzazione della manovra stessa. È palese che, nel caso in oggetto, abbiamo di fronte a noi un provvedimento collegato i cui contenuti vanno ben al di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF votata a luglio. Peraltro, alcuni articoli del provvedimento originario - volti a tipizzarne il suo contenuto, prettamente di carattere finanziario - sono stati da esso espunti e trasposti in altri provvedimenti già approvati dal Parlamento.

lo pone insomma lontano dal configurare qualsiasi politica di settore equilibrata e completa. La drammatica attuale situazione del lavoro in Italia, caratterizzata, come già ben illustrato dal collega Lannutti, dalla presenza di un vero e proprio esercito di lavoratori precari richiedeva e richiede ben altro approccio e ben altre soluzioni. Noi non possiamo che ribadire la nostra preoccupazione. Il nostro Paese si sta avviando, secondo previsioni sia nazionali che internazionali, verso la quota di 500.000 lavoratori disoccupati in più, verso quella situazione, lo ribadiamo ancora, di crescita senza occupazione che rischia seriamente di lasciare una pesante eredità sociale per gli anni a venire. Non ci sembra davvero che con tali norme si possa contribuire ad affrontare seriamente questa drammatica

prenderò la parola per qualche minuto per ribadire l'importanza del disegno di legge su cui fra poco saremo chiamati al voto finale, in un'Aula desolatamente vuota, e questo deve farci riflettere. Questo testo, infatti, scaturito da un lungo percorso di confronto e da modifiche apportate in sede di Commissioni riunite e di Aula, contiene importanti misure in tema di lavoro sia privato che pubblico. Di primaria importanza è la revisione del processo del lavoro, in particolare per quanto riguarda il ricorso alla conciliazione, non più obbligatoria prima dell'apertura di una causa davanti al giudice, così come previsto da alcune proposte emendative presentate alle Commissioni di merito dal Gruppo Lega Nord. Siamo inoltre soddisfatti per l'approvazione in quest'Aula degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo che riguardano le organizzazioni sindacali ed introducono il criterio ragionevole della rappresentatività a livello di amministrazione o su base territoriale, dando in questo modo maggior forza alla rappresentanza degli interessi dei nostri lavoratori.

che impegna il Governo a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti pubblici, ovvero che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici. Inoltre, nel testo dell'ordine del giorno viene previsto che il Governo debba riferire al Parlamento tutti i casi in cui il compenso di questi managersuperi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Bisogna tagliare quei privilegi di cui godono i super manager. Non si può più accettare lo spreco di risorse pubbliche per pagare stipendi d'oro a dette persone. Questa maggioranza dall'inizio della legislatura ha dimostrato ampia sensibilità nei confronti delle problematiche lavorative. Vorrei ricordare a tal proposito il varo del cosiddetto decreto Brunetta sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sull'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Diverse norme contenute inizialmente nel collegato in esame sono state inserite nella riforma Brunetta. Una su tutte che mi preme ricordare, e che è stata fortemente voluta e sostenuta dal Gruppo Lega Nord, è quella riguardante la territorializzazione dei concorsi pubblici, *ex* articolo 6 del testo in esame, ed ora contenuta in uno dei decreti legislativi attuativi della legge Brunetta. Nella proposta di legge che quest'Aula sta ora esaminando sono comunque contenute altre norme sul lavoro pubblico, le quali vanno sempre nella direzione di attuare politiche di rinnovamento volte a risolvere i problemi di inefficienza e di inefficacia dell'attuale pubblica amministrazione. Per fare ciò, ci si attende che il mercato del lavoro pubblico converga verso quello del lavoro privato, anche prevedendo forme di mobilità del personale e rendendo trasparenti le valutazioni dell'operato degli addetti alle funzioni pubbliche. Vengono inoltre previste misure atte a garantire pari opportunità ed assenza di discriminazione nelle pubbliche amministrazioni. Questa coalizione di Governo sta facendo molto per la nostra gente e sta adottando provvedimenti importanti in tema di lavoro e anche in tema di sicurezza sul lavoro. prima della pausa estiva, è stato portato a compimento il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (e anche in quel caso, ricordo, in un'Aula desolatamente vuota). un segnale di come l'attuale maggioranza abbia una intenzione specifica nella risoluzione definitiva di questo grave problema, che comunque non ha e non può avere un colore politico. Infatti, ogni giorno si apprendono notizie riguardanti lavoratori che perdono la vita o rimangono feriti gravemente mentre svolgono il loro lavoro. Questa realtà sta determinando una vera e propria emergenza sociale, una guerra silenziosa, che deve richiamare tutti, e le e le istituzioni per prime, ad intervenire per regolare con maggiore e assiduo impegno un mercato del lavoro non sempre rispettoso delle regole e spesso indifferente alla tutela fisica dei lavoratori. È soprattutto nell'economia sommersa che si verifica il maggiore numero di morti bianche. Nel disegno di legge che stiamo per votare oggi, in questa Assemblea, si definiscono nuove misure contro il lavoro sommerso, un fenomeno da contrastare con ogni mezzo, fuori da ogni regola basata sull'utilizzo e lo sfruttamento per lo più della manodopera extracomunitaria irregolare. È proprio qui che si verificano commistioni tra il cosiddetto lavoro nero e l'immigrazione clandestina. All'interno di questo quadro già complesso della condivisione del lavoro nel nostro Paese si aggiunge sfortunatamente anche il basso potere d'acquisto degli stipendi e dei salari della nostra gente che, nel momento economico attuale, non riesce ad arrivare con tranquillità alla fine del mese e che cerca di far fronte alle cresciute difficoltà economiche ricorrendo al cosiddetto doppio lavoro. È necessario quindi, e non più rinviabile, un intervento per garantire ai nostri lavoratori un potere di acquisto che non vada via via diminuendo, come sta accadendo in questi ultimi tempi. Siamo di fronte ad una realtà in cui c'è un forte freno allo sviluppo del Paese, che mette in seria difficoltà le famiglie, che non ce la fanno ad arrivare alla terza, e a volte alla seconda settimana del mese. Questo - lo ribadisco - è un tema reale che deve essere affrontato in tempi brevi. Siamo soddisfatti dell'approvazione dell'ordine del giorno che impegna il Governo a valutare, in sede di presentazione degli atti di indirizzo per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, nel limite delle risorse stanziate, l'applicazione di un coefficiente del territorio utile per la rivalutazione delle retribuzioni e degli stipendi pubblici che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale. Vorrei ricordare che vi sono state ragioni storiche e sociali, che hanno caratterizzato gli anni Cinquanta e Sessanta, che hanno portato all'approvazione dello Statuto dei lavoratori e ad una retribuzione uguale ed uniforme per tutti. A quarant'anni di distanza dall'introduzione del sistema di contrattazione collettiva su base nazionale e dopo l'abolizione della scala mobile - vorrei ricordarlo ai miei colleghi senatori *ex* sindacalisti non vi sono però stati altri elementi regolari che abbiano mantenuto il rapporto stipendi‑costo della vita in equilibrio o che abbiano cercato di porre rimedio alle differenze economiche che permangono nelle diverse realtà territoriali. Con l'intento di garantire uguali diritti a tutti i lavoratori, si è creato invece un sistema che ha fatto aumentare la disparità tra loro. Se è vero che in questo contesto certe politiche avevano un senso, in quello attuale sono assolutamente inadeguate e obsolete, e quindi, ora quanto mai, è necessario promuovere una riforma del sistema che, nel rispetto dei diritti acquisiti, segua i princìpi costituzionali dell'uguaglianza sostanziale e del diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa. La Lega Nord Padania vuole intervenire in maniera decisa per non deludere coloro che hanno dato la loro fiducia alle nostre battaglie ventennali e dare finalmente quelle risposte che la nostra gente si aspetta. È necessario introdurre un principio per l'applicazione di un coefficiente del territorio per la rivalutazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, nella convinzione che possa servire da esempio e da volano per una riforma in senso territoriale della contrattazione anche nel settore privato. Anche un maestro delle riforme in tema di lavoro, come Marco Biagi, nel Libro bianco sul lavoro rilevava, tra l'altro, che ciò che deve essere salvaguardato non è non è tanto il valore assoluto della retribuzione, bensì il suo reale potere di acquisto. In questa idea vi era una spinta sociale e riformatrice, propensa al cambiamento, in cui noi, come Lega Nord, ci riconosciamo in pieno. Mi auguro che quest'Aula possa cogliere il significato più profondo delle mie parole e capisca quanto ormai sia arrivato il momento di attuare un'importante riforma del mercato del lavoro per una nuova società, moderna e al passo con i tempi. Come Gruppo Lega Nord, non ci stancheremo mai di ripetere che questo Paese ha bisogno delle riforme. Per noi è diventato un obbligo morale: in campagna elettorale abbiamo fatto delle promesse, e ora, con i fatti e il nostro impegno, le porteremo avanti. L'attuale maggioranza ha già intrapreso un percorso di riforme

politiche, sindacali, datoriali e alle banche. Bisogna andare avanti con il processo riformista attraverso un confronto costruttivo, fuori dagli schemi ideologici e di contrapposizione tra i diversi schieramenti. Occorre evitare strumentalizzazioni, che non servono certo per risolvere i problemi del Paese. Bisogna cercare invece di fornire risposte concrete al mondo del lavoro e alle imprese, che si trovano in un periodo di difficoltà. Le riforme vanno assolutamente affrontate senza pregiudizi e senza esasperare gli scontri o i toni del dibattito, seguendo la strada del dialogo, che da sempre vogliamo percorrere. Gli interessi dei lavoratori non sono mai parsi in conflitto con l'interesse della crescita e dello sviluppo dell'intero Paese. Ci auguriamo, quindi, che questo provvedimento e tutti gli interventi posti in essere dalle istituzioni per rinnovare il mondo del lavoro possano essere attuati concretamente e possano produrre quei risultati da tempo auspicati. Quarant'anni fa, in occasione dello sbarco sulla luna, si parlò di questo evento come di un piccolo passo per l'uomo, ma di un balzo gigantesco per l'umanità. Speriamo che l'approvazione dell'ordine del giorno in tema di riforma delle buste paga in senso territoriale sia un piccolo passo che possa portare ad un importante miglioramento della vita di tutti i giorni della nostra gente. Per queste ragioni, esprimo, a nome del Gruppo che qui rappresento, il voto favorevole della Lega Nord sul disegno di legge in esame.

a vedere dei segnali di ripresa. Per fare questo, non occorrono provvedimenti tampone, disorganici, come sono in larga parte questi, ma

dell'intermediazione a titolo gratuito, e dunque un doveroso richiamo a regole internazionali, è stata incomprensibilmente espunta. Ciò ha a che fare anche con la confusione in cui si è

irregolari, e abbiamo apprezzato qualche norma sulla trasparenza nel pubblico impiego, che è una vecchia battaglia che abbiamo condotto anche in altra sede. qualcuno di questi provvedimenti è anche merito nostro, ma si perde nel *mare magnum* di questo contenitore indistinto. nel merito interventi gravi, che indicano una linea di tendenza che potenzialmente non è di flessibilizzazione razionale dei mercati, del lavoro e dei servizi, ma di deregolazione sconsiderata. insieme a interventi che con un po' di velleitarismo vorrebbero raddrizzare le gambe a punti specifici, per esempio in materia di pubblico impiego, che richiederebbero ben altri interventi.

cosa vogliamo fare? Mettiamo insieme due o tre organismi che non ci azzeccano niente - come si suol dire - con il risultato di indebolire ulteriormente un settore critico. Questi, quindi, specifici molto negativi, che indicano una linea di tendenza sbagliata, i più gravi dei quali - come abbiamo segnalato - riguardano proprio il cuore del diritto del lavoro. Le critiche che abbiamo mosso alle norme sulla certificazione e sull'arbitrato

proposta non è stata accettata, si passa all'estremo opposto, per cui siamo l'unico Paese del mondo che fino a ieri non aveva l'arbitrato in materia di lavoro e oggi ne ha uno libero per iniziative individuali, cosa che non esiste neanche in Uzbekistan.

ho esemplificato alcuni punti che dimostrano che abbiamo perso un'occasione per aiutare, anche con questo provvedimento, la ripresa. Vi abbiamo inserito delle zeppe

e che, dopo l'acquisizione delle riflessioni e delle opinioni delle organizzazioni sindacali e datoriali, nonché degli enti, delle associazioni e degli istituti di ricerca interessati, si è protratto per 21 sedute. Le numerosissime modifiche al testo giunto dalla Camera sono state accolte in seguito alla presentazione di più di 400 emendamenti, principalmente d'iniziativa parlamentare. Essendosi l'esame del testo protratto per un periodo assai ampio, è ovvio che al contempo siano intervenuti vari provvedimenti che il Governo ha posto in essere, con carattere di urgenza, al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale, sostenere il reddito dei lavoratori e promuovere la ripresa degli investimenti e dei consumi. Le modifiche introdotte al testo originario hanno dunque avuto anche lo scopo di adeguare il testo alle disposizioni legislative nel frattempo intervenute. Nel complesso, il disegno di legge reca - in parallelo rispetto agli interventi urgenti già effettuati - un'opera più meditata di modifica di alcuni istituti giuridici del mercato del lavoro e del processo del lavoro. Al riguardo si tratta peraltro solo di un primo passo, in quanto il provvedimento reca diverse deleghe, oltre a riaprire i termini di alcune deleghe scadute. Tale è il caso delle deleghe concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile, che richiederanno sicuramente un'opera di riscrittura di diverse parti della legislazione in materia di lavoro adottata negli ultimi decenni. In particolare, il tema dell'occupazione femminile - è bene ricordarlo e sottolinearlo - costituisce uno dei problemi principali che deve affrontare il nostro Paese ai fini della della crescita del tasso di occupazione e del prodotto interno e, quindi, anche ai fini della sostenibilità finanziaria, nei prossimi decenni, nonché del costo crescente dei sistemi di previdenza sociale e di sanità pubblica. Non mi soffermo sugli aspetti riguardanti il mondo del lavoro nel pubblico impiego, che hanno subito anch'essi delle modifiche: il nostro intervento legislativo si è infatti conformato conformato nel tempo alla riforma attuata dal ministro Brunetta, che, attraverso il decreto legislativo n. 150 del 2009, ha voluto imprimere un segno concreto di efficienza e modernizzazione del nostro apparato amministrativo per renderlo rispondente ai principi di sussidiarietà e responsabilità nell'erogazione dei servizi offerti ai cittadini. Riguardo alle norme immediatamente precettive, desidero però sottolineare le modifiche apportate al cosiddetto decreto Biagi: si tratta, infatti, di modifiche importanti che, nel muoversi nella filosofia di fondo di quel decreto, ne completano però il disegno. Un particolare rilievo assume in questo quadro la reintroduzione della possibilità di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto *staff leasing,* uno strumento prezioso che verrà così posto a disposizione soprattutto delle piccole imprese, consentendo loro di accedere a qualificati strumenti gestionali in modo congiunturale, senza doverne pagare gli alti costi operativi. In conclusione, la struttura del provvedimento, basata sul ricorso alla delega legislativa, appare pienamente motivata dalla complessità e dalla difficoltà di gran parte della materia cui esso attiene. Ciò permetterà di intervenire, nell'ambito di principi e criteri direttivi fìssati dal Parlamento nelle deleghe stesse, in modo mirato ed efficace, con l'adeguata e necessaria duttilità. Complessivamente, il provvedimento rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto già contenuto nella cosiddetta legge Biagi, di cui costituisce una conferma ed un completamento al tempo stesso, e presenta punti di forza particolari che costituiscono la traduzione concreta di alcuni impegni qualificanti assunti nel programma di Governo. I dati recentemente elaborati e resi noti dall'OCSE hanno confermato che, rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia ha saputo affrontare la crisi complessiva con strumenti dotati di una più spiccata capacità di incisione e che dunque essa prima e meglio degli altri si sta avviando verso una fase di segno positivo. Proprio alla stregua di queste considerazioni va letto quel capitolo del provvedimento che si riferisce agli ammortizzatori sociali: un tema, questo, sul quale il Governo si è mosso con tutta la duttilità necessitata dall'alluvionalità della crisi che ha colpito il nostro Paese, Paese, resa ancora più drammatica dallo scenario devastato dell'intero panorama economico-finanziario del mondo globalizzato. Il testo assume un particolare rilievo per tutta la parte che rivisita il processo del lavoro, con una particolare enfasi sul ruolo della conciliazione e dell'arbitrato, che accentua e valorizza l'autonomia delle parti contrattuali e sociali. A questo riguardo, a proposito delle osservazioni mosse dal senatore Treu, non posso che rimandare a quanto già osservato in tema di intervento su quell'articolo: il principio dell'autonomia privata, che è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema civilistico, è stato riaffermato in maniera certa: principio dell'autonomia contrattuale che fa parte del concetto di libertà inteso in senso ampio e che non conosce limiti, se non quelli che indica lo stesso codice, laddove si parla di autonomia privata che comunque non collida con le norme imperative, con le norme relative all'ordine pubblico e al buon costume. Al di fuori di questi limiti posti dal nostro sistema, l'autonomia contrattuale può espandersi nel modo che più si crede opportuno. Abbiamo dato voce a questo principio fondamentale, e abbiamo fissato alcuni paletti, per evitare che interpretazioni, sicuramente non condivisibili o per lo meno conflittuali, potessero andare contro il bene fondamentale della chiarezza e della certezza del diritto. È questo un tema fondamentale sul quale, più che ricevere i moniti del centrosinistra, preferiamo prenderci i meriti di questa coraggiosa riforma effettuata.

se non addirittura dirompente: si degiurisdizionalizza, in questo modo, un processo la cui introduzione, come ben sanno gli operatori e gli studiosi, fu motivata dall'esigenza di garantire celerità ed immediatezza, e che a maggior ragione necessita oggi di tempi rapidi.

si configurano in linea con gli obiettivi preannunciati dal ministro Sacconi all'interno del Libro verde sul futuro del modello sociale. Il *target* imposto dal Trattato di Lisbona (tasso di occupazione al 70 per cento, con un 60 per cento di occupazione femminile) deve infatti essere inteso come un obiettivo concreto che si realizza solo con la partecipazione dei cittadini ad un mercato del lavoro regolare, che é il primo passo verso la «vita buona» di cui si fa menzione nel Libro bianco. Sono queste le ragioni che spingono il nostro Gruppo a sostenere questo provvedimento.

per un sistema che sicuramente riceve una profonda innovazione, ciò che è il primo passo verso la strada così icasticamente disegnata nel Libro bianco del ministro Sacconi.

Il relatore, senatore Bettamio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

non solo perché essi costituiscono uno dei principali mercati per l'esportazione di materiale di armamento italiano, ma anche perché sono il principale mercato mercato di sbocco delle nostre esportazioni in Medio Oriente e in Nord Africa. Se le mie informazioni sono esatte, abbiamo superato, per quanto riguarda il saldo delle esportazioni, il tradizionale partner commerciale degli Emirati, che è la Francia. Ciò vale anche per la presenza dei nostri imprenditori, che in quello Stato

come ricorderanno i colleghi senatori, questo Accordo aveva presentato una serie di criticità nel suo primo passaggio al

Nel passaggio alla Camera dei deputati, alcune di queste criticità sono state prese in considerazione, tanto è vero che è stato aggiunto l'articolo 3 in cui si prevede che: «Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni». dell'Accordo «al fine di semplificare l'attuazione delle procedure concernenti la supervisione delle attività di importazione ed esportazione di mezzi e materiali d'armamento» non aveva previsto questo meccanismo. Secondo l'opposizione, tale mancanza era particolarmente grave perché, se andiamo a vedere

Auspichiamo, quindi, pur mantenendo il nostro parere, a questo punto in parte risolto dalla modifica ottenuta alla Camera, che si possa includere all'interno dell'avvio dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti

tra le varie attività che godranno della cooperazione sviluppata tra le parti, vi sono anche le attività culturali e sportive in campo militare.

Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, dobbiamo avere molta cura di non considerare queste ratifiche delle sinecure, per l'appunto, o degli atti strettamente burocratici.

poi per quanto può essere implicito in stesure così vaghe e onnicomprensive. Materiali specifici per uso militare: cosa sono?

non risulta che ci sia stata questa visione catastrofista in Commissione esteri quando si è esaminato il provvedimento. è un rapporto di collaborazione sulle politiche della difesa, un'operazione sempre nel settore della difesa, ed è vero che è anche un rapporto sul fronte della eventuale fornitura di armi o di armamenti. Ricordiamo che noi abbiamo soldati presenti su scenari diversi, tra cui l'Afghanistan, che non è raggiungibile con mezzi civili.

oltre a produrre tante altre cose, l'Italia ha un'industria bellica importante che produce elicotteri appetibili e ha stipulato una convenzione prima con gli *Eurofighter* e poi con gli JSF che saranno i prossimi aerei, costruiti in parte anche in Italia, che adotteranno tutte le aeronautiche dei Paesi più sviluppati. Ebbene, guardiamo anche a questo settore con una certa attenzione e non con noncuranza o addirittura con una preoccupazione aprioristica e ingiustificata. Gli Emirati sono l'unica finestra dell'Europa sull'Asia. Oggi abbiamo degli ottimi rapporti e il mio intervento, più che rispondere ai colleghi, era mirato a proporre un'osservazione al sottosegretario Mantica. Gli Emirati hanno una forte volontà di collaborare con l'Europa e in particolare con l'Italia. Infatti collaborano con i nostri militari, ma si sentono un tantino

questo Accordo ritorna per la ratifica, come ha ricordato il collega Perduca, dopo una discussione alla Camera

ma, a meno che non vi sia un'obiezione generale a qualsiasi accordo che riguardi la cooperazione nel campo della difesa, e che quindi riguardi naturalmente la fornitura di armi e di apparati militari, non è francamente data, a mio parere, una ragione per cui accordi di questo tipo possano essere conclusi con altri Paesi e non con gli Emirati Arabi Uniti. Non esiste una ragione specifica che si possa opporre:

esteri*. Signor Presidente, credo che il dibattito abbia assolutamente chiarito le ragioni per cui il Governo porta in Aula la ratifica. Si è discusso molto; il Governo ha accettato alla Camera di fare un emendamento che noi crediamo garantisca - come peraltro lo stesso senatore Perduca ha riconosciuto - alcune garanzie nella gestione di questo accordo. Il Governo in questa sede non può che sottolineare l'urgenza e l'importanza strategica di un accordo di questo tipo con gli Emirati Arabi Uniti.

Signor Presidente, pur votando favorevolmente, continuiamo ad avanzare la legittima pretesa che in futuro si provveda ad eliminare del tutto il termine mine da questo accordo stipulato con gli Emirati Arabi e nel prosieguo. Mi vedrà altrimenti costretto a non votare più le ratifiche internazionali per quello che riguarda l'inserimento di questa parola. Cari colleghi, ci troviamo anche oggi a votare su disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. L'argomento delle ratifiche è trattato, come spesso ho denunciato, alla stregua di un tappabuchi - lo ha detto anche il collega Perduca - per quei momenti in cui la Presidenza non sa cosa mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato. Noi dell'Italia dei Valori ci siamo sempre opposti a questa concezione della politica estera da parte dell'Assemblea parlamentare, come di una burocratica ratifica di accordi stretti dal Governo, sulla quale il Parlamento non abbia niente da dire a da modificare con la sua riflessione. Ho denunciato la scarsa partecipazione dei colleghi, i pochi interventi e la mancanza di dibattito. Forse appunto per questo condivido la tesi del collega Perduca di chiedere il voto elettronico in futuro se non

PdL)*. Ho denunciato questa scarsa partecipazione, ma oggi devo dirvi che al disinteresse del Parlamento non posso che dare ragione. È ormai chiaro, infatti, che il Parlamento di politica estera non può occuparsi in questa legislatura. Questo paradigma allarmante ce lo ha chiarito ieri sera il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il Presidente del Consiglio, infatti, alle ore 18,25 di ieri ha diramato un comunicato stampa nel quale ha affermato: «Ho ricevuto una telefonata da parte del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nel corso della cordiale conversazione è stata esaminata principalmente la situazione in Afghanistan ed il Presidente americano ha illustrato i punti salienti della revisione strategica che l'amministrazione Usa Usa si appresta a varare. Il presidente Obama ha elogiato il ruolo di *leadership* svolto dal presidente Berlusconi sulla questione afgana e sui numerosi altri teatri di crisi, chiedendo il sostegno dell'Italia nel rafforzamento dell'impegno della comunità internazionale in Afghanistan. Il *Premier* ha accolto positivamente questa richiesta». Questo è ciò che abbiamo letto, cari colleghi. Ebbene, io trovo che sia raccapricciante che Berlusconi decida, da solo, sul potenziamento dei soldati italiani in Afghanistan

Io trovo che sia raccapricciante che ciò avvenga mentre il disegno di legge di proroga delle missioni è ancora in discussione davanti alle Commissioni riunite Trovo raccapricciante che Berlusconi faccia promesse di inviare soldati in Afghanistan, quando in finanziaria i soldi per le missioni internazionali non ci sono. Non ci sono! *(Proteste dal

indirettamente li stimola. PEDICA *(IdV)*. Voi continuate a votare anche se non ci sono i soldi. L'annuncio di Berlusconi mi ricorda tanto quello fatto da un altro *leader* italiano il 10 giugno del 1940 dal balcone di Piazza Venezia,

Anche allora non c'erano i soldi per garantire sicurezza ai soldati, che andavano in guerra con le scarpe di cartone. Anche allora i cittadini non venivano consultati in merito alla missione, come oggi il Parlamento non viene ascoltato sull'Afghanistan, o si promette di farlo solo dopo l'annuncio, per rimediare all'ondata di dissenso. Anche allora si smarriva il senso dei valori italiani per compiacere qualche *leader* straniero. Ecco perché il comunicato stampa del presidente del Consiglio Berlusconi di ieri mi ha totalmente convinto del fatto che il Parlamento in questa legislatura non si occupa e non si occuperà mai di politica estera. Ecco perché adesso capisco il disinteresse alle ratifiche dei trattati internazionali, contro il quale mi ero ingiustamente opposto in questi mesi. Ecco perché non interverrò per nessuna dichiarazione di voto ma consegnerò ogni mio intervento. per protesta contro una politica estera dittatoriale e antidemocratica, per protesta contro il mancato coinvolgimento del Parlamento su un tema delicatissimo come quello dell'Afghanistan, sul quale la posizione dell'Italia dei Valori è dolorosamente attenta alla situazione dei militari e alle finalità di pace delle missioni, ed è assolutamente convinta che quella in Afghanistan abbia ormai mutato natura, divenendo una missione di guerra. Il 2009 ha registrato una *escalation* di guerra dichiarata, sia per il livello di conflittualità dei talebani che per il numero di vittime, più di 400 da gennaio solo fra i soldati stranieri. Lo annuncio già da oggi, cari colleghi: l'Italia dei Valori voterà no all'articolo sull'Afghanistan inserito nel decreto di proroga delle missioni in discussione al Senato, e si asterrà sul provvedimento nel complesso. infatti convinti che la presenza italiana in quell'area non è più rispondente alla finalità di ricostruzione con la quale la missione è iniziata nel 2004. C'è infatti una forte contraddizione fra la missione e i nostri valori costituzionali. *(Commenti dal Gruppo PdL).* Abbiamo presentato un emendamento al decreto di proroga delle missioni con il quale chiediamo di concordare multilateralmente presso ONU e NATO una *exit strategy* da finalizzare entro febbraio prossimo. Ma dopo la telefonata di Berlusconi,

che di fronte a tale gesto unilaterale di Berlusconi sul dossier più caldo della nostra politica estera, ossia l'Afghanistan, sulle ratifiche di accordi con Panama o con la Romania non ritengo ormai più logico impegnare il tempo mio e quello dei colleghi. Ecco perché consegnerò il testo dei miei interventi. Ecco perché l'Italia dei Valori a questo sistema di condurre la politica estera non ci sta.

annunzio soltanto il mio voto favorevole, per le ragioni esposte dal relatore e per quelle richiamate dal sottosegretario Mantica, nonché per quelle illustrate dal collega Marcenaro. Gli altri argomenti mi sembrano un po' estranei all'ordine del giorno di oggi.